«Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico» (1272). In data 19 ottobre 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze: «Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» (1274).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

In Polonia l’aborto è permesso solo in caso di incesto, stupro o pericolo di vita per la donna. Fino al 2020 era consentito anche in casi di gravi malformazioni del feto, ma il 22 ottobre di quell’anno la Corte costituzionale polacca ha eliminato questa possibilità. settembre 2021 una donna polacca di trent’anni è morta di shock setticemico perché i medici, a causa proprio delle restrizioni imposte dalla legge, non le praticarono l’aborto terapeutico, aspettando invece che morisse il feto. Lo scorso dicembre la Corte europea dei diritti umani (CEDU) ha stabilito che la sentenza della Corte polacca viola l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti Anche in Italia il diritto all’aborto sta subendo un attacco concentrico. L’ultima relazione del Ministero della salute sull’applicazione della legge n. 194 del 1978 dimostra, dai dati ministeriali, che in Abruzzo, in Molise e in Sicilia i medici obiettori sono quasi nove su dieci, mentre in Campania, Puglia e Basilicata sono otto su dieci. Inoltre, l’aborto farmacologico è osteggiato e, anche laddove l’interruzione volontaria di gravidanza è praticata, le donne sono spesso oggetto di commenti, domande e comportamenti inappropriati che rendono l’aborto un’esperienza psicologicamente violenta. Tutto ciò mentre le organizzazioni antiabortiste sono finanziate coi soldi pubblici per molestare le donne anche all’interno degli stessi consultori. Nell’Europa dei diritti ciò non è più tollerabile. È per questo che, come MoVimento 5 Stelle, insieme all’Alleanza Verdi e Sinistra, sosteniamo con convinzione l’iniziativa «My voice my choice» per arrivare entro dicembre a un milione di firme e spingere il Parlamento europeo

Signora Presidente, a nome del Partito Democratico mi associo alle istanze rappresentate dalla collega nell’anniversario della sentenza polacca contro l’aborto e contro le donne e i loro corpi.

dicevo che mi associo alle istanze rappresentate sulla sentenza polacca contro l’aborto, contro le donne, i loro corpi, la loro libertà in Polonia, come in ogni Paese in cui questo diritto viene posto in discussione, diminuito, messo a repentaglio a lei, signora Presidente, e all’Assemblea che poche ore fa, nell’ambito di uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, è stato liberato Oleksiy Bura, uno dei difensori di Azovstal, le Termopili di Mariupol. Catturato, portato in Russia, processato per direttissima, condannato all’ergastolo solo per aver difeso la sua città, Oleksiy, in carcere da due anni, è gravemente malato. Racconto brevemente la storia di questo ragazzo ucraino che, come tanti, ha resistito alla spietata invasione russa, perché sua moglie Vialyetta, una studentessa di ventitré anni, la scorsa estate è venuta proprio qui in Senato, assieme ad altre tre donne (Alla, Tamara e Tetyana), madri e mogli di prigionieri di guerra, soldati condannati a pene a vita, detenuti nelle infernali carceri artiche, le stesse dov’era rinchiuso ed è stato ucciso Aleksej Aleksej Navalny. Queste donne hanno fatto il giro del mondo per sensibilizzare parlamenti e opinione pubblica sulle sorti dei loro congiunti, disperata speranza. Hanno incontrato anche il Papa e voglio pensare che proprio questa intercessione - la scorsa settimana il cardinale Matteo Zuppi è stato in Russia - sia stata preziosa, perché finalmente la scorsa notte Oleksiy ha potuto riabbracciare sua moglie. Credo che il sostegno risoluto politico, economico e militare del nostro Paese all’Ucraina, alla difesa della democrazia e delle libertà, sia un dovere ineludibile e resistente, così come l’azione diplomatica ad ogni livello, perché l’aggressione russa possa terminare ed essere respinta e uomini come Oleksiy, il cui unico crimine è stato quello di

alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno: Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari La seduta è tolta